dal più alto scranno istituzionale della nostra Repubblica, è venuto un invito ad una distensione dei toni delle polemiche.

veicolato ai cittadini e che nessuno si è premurato di smentire. A questa cena avrebbero

Corte costituzionale avrebbe preparato per modificare la Costituzione nella parte riguardante la magistratura. Si tratta di interrogativi di particolare rilievo e di notevole gravità, che imporrebbero al Ministro della giustizia di rassicurare il Parlamento e il Paese sui contenuti di questa cena, se mai si è verificata.

ovviamente non entrerò nel merito di tutte le questioni sollevate ieri dai colleghi di opposizione nelle loro numerose questioni pregiudiziali, perché non ne avrei il tempo.

e abbiamo analizzato, anche vivacemente, tutti gli elementi sollevati ancora ieri nelle questioni pregiudiziali. Pertanto, non mi soffermerò sui temi della sicurezza partecipata, delle ronde, dell'accesso ai pubblici servizi da parte dei clandestini,

è praticamente la fotocopia di due pareri espressi dal Consiglio superiore della magistratura sul decreto-legge in materia di violenza sessuale

Il contenuto testuale dei due pareri è stato riportato all'interno di questa questione pregiudiziale, per cui oggi abbiamo anche l'anomalia parlamentare ‑ e, credo, istituzionale ‑ di doverci pronunciare su una questione pregiudiziale che riporta testualmente il contenuto -

sia una pagina felice delle istituzioni parlamentari, e forse può far riflettere anche sul ruolo del CSM e sul suo compito di esprimere giudizi ‑ purtroppo di natura politica, e di politica criminale ‑ sulle leggi che adottiamo. Mi soffermerò, invece, sul punto relativo al reato di clandestinità, sul quale forse si sono sentiti elementi nuovi. Per la verità, il nuovo elemento di chiarezza è venuto dalla dichiarazione di voto svolta alla Camera dal segretario del Partito Democratico Franceschini, quale ha detto con estrema chiarezza che con il reato di clandestinità e l'aggravante della clandestinità si colpisce lo straniero non per quello che ha fatto, ma per quello che è e per la storia che ha.

l'appello dei cosiddetti giuristi contro il reato di immigrazione clandestina pubblicato pochi giorni fa riporta una posizione culturale identica. In sostanza, si dice - e ne riporto le testuali «l'ingresso o la presenza illegale del singolo straniero dunque non rappresentano, di per sé, fatti lesivi di beni meritevoli di tutela penale, ma sono l'espressione di una condizione individuale, la condizione di migrante». il disvalore e l'offensività della condotta di uno straniero che entra illegalmente in questo Paese, senza rispettare le regole d'ingresso fissate dal nostro Parlamento e in totale spregio delle nostre frontiere, o che vi risiede illegalmente, senza rispettare le regole di soggiorno, esiste o non esiste? Secondo la vostra posizione culturale sostanzialmente non esistono alcun disvalore e alcuna offensività nella condotta di uno straniero che non rispetta le regole d'ingresso e di soggiorno di questo Stato. Non c'è per voi nessun disvalore, perché queste sono espressioni della condizione di migrante.

E la condizione di migrante, secondo la vostra posizione culturale, autorizza la violazione delle frontiere, quasi vi fosse una sorta di libera circolazione del clandestino che può varcare le frontiere di questo Paese senza alcun rispetto per le regole di controllo dell'immigrazione. Anzi, mentre lo straniero regolare non ha un diritto soggettivo a entrare in questo Paese, ma può presentare una domanda che viene vagliata dalle autorità di pubblica sicurezza, il clandestino migrante ha un diritto soggettivo a entrare e uscire da questo Paese a suo piacimento.

vi ricordo solo una cosa, colleghi, anche perché abbiamo stima di molti di voi: la posizione culturale che porta alle conseguenze politiche che avete illustrato ieri è pericolosa perché mina le fondamenta di questo Stato. Ed è un paradosso che la forza, il movimento meno statalista in questo Parlamento debba cercare di evidenziare tale aspetto, perché l'ente Stato è composto da tre elementi costitutivi: un governo, un popolo ed un territorio.

sulla quale occorre dare risposte convincenti per contrastare in maniera inflessibile il fenomeno dell'immigrazione irregolare e per combattere la clandestinità. Ripeto, sto usando il verbo impiegato nel Patto europeo sull'immigrazione dell'ottobre 2008: il Consiglio europeo ci chiede di combattere l'immigrazione clandestina,

dei beni e dei delicati interessi in gioco: da un lato, il principio di uguaglianza e l'offensività che voi richiamate spesso, dall'altro anche il principio della sicurezza e della libertà personale, soprattutto delle persone più deboli.

che, nello sviluppo dei sistemi costituzionali moderni, l'idea e il principio di libertà e di democrazia

nella nostra Costituzione, ma anche e soprattutto nei provvedimenti di diritto e delle convenzioni internazionali, a partire dalla Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo del 1948. Questi princìpi si radicano, ancor più, nel lungo viaggio del costituzionalismo occidentale e, addirittura, nella *Magna Charta* del 1215: anche allora, accanto all'idea di libertà, veniva annotato il diritto alla sicurezza. Per entrare nel merito delle eccezioni che sono state qui prospettate e, quindi, per delineare l'ambito degli interventi, vorrei aggiungere anche

una legge costituzionale che può essere interpretata - come hanno fatto alcuni colleghi dell'opposizione - in modo sistematico come se fosse, appunto, una legge ordinaria. sviluppa e garantisce dei principi fondamentali e dei diritti di libertà. Il quadro dei diritti fondamentali deve essere appunto legato allo sviluppo storico di questi diritti di libertà.

evocati, la censura alla norma che introduce il diritto dei cittadini di fondare associazioni finalizzate a segnalare alle Forze di polizia statali e locali eventi che possano arrecare danni alla sicurezza urbana e alla coesione sociale. vorrei qui ricordare che la Costituzione del nostro Paese, all'articolo 18, garantisce e tutela il diritto di associazione dei cittadini;

vietano tre tipi di associazioni: quelle vietate dal codice penale in quanto il fatto di associarsi costituisce ipotesi di reato; la norma contenuta nelle disposizioni di attuazione della Costituzione, cioè il divieto di associazioni con il fine di ricostituire il partito fascista; il divieto di associazione di carattere militare e di fondare associazioni di carattere segreto. fatta eccezione per questi tre tipi di associazioni, in questo momento, se non si introducesse una norma che ne regola e ne dettaglia la disciplina, qualunque cittadino o gruppo di cittadini potrebbe fondare un'associazione con il fine, appunto, di realizzare ciò che la norma invece introduce.

quale la Repubblica riconosce e garantisce non solo i diritti inviolabili dell'uomo, ma soprattutto quelli che si sviluppano nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Pertanto le associazioni sono lo strumento principale per la realizzazione e la partecipazione dei cittadini a quel dovere di solidarietà sociale richiamato sempre dall'articolo 2. 2. Se questa non fosse la base attraverso cui le associazioni si muovono, dovremmo sostenere che anche la disposizione contenuta nel codice penale in forza della quale i cittadini hanno l'obbligo di denunciare fatti di reato contro la personalità dello Stato Stato puniti con la pena dell'ergastolo sarebbe in palese violazione della Costituzione. Così come, sulla base delle tesi prospettate, sarebbe incostituzionale la norma che prevede la facoltà di arresto in flagranza di reato in capo ai cittadini. In realtà, queste disposizioni sottolineano l'esigenza di rafforzare la partecipazione dei cittadini alla tutela degli interessi generali e corroborano in modo particolare il civismo, il senso civico dei cittadini italiani. Quindi, non c'è alcun profilo di incostituzionalità della norma

delle norme del soggiorno era già presente nel nostro ordinamento già dall'introduzione del primo Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con la legge del 1865, n. 2248, allegato B.

poi enucleata e depenalizzata con la riforma del ministro Martelli del 1988. Ebbene, l'incongruenza in cui incorre l'ordinamento - e per questa ragione intendiamo colmare la lacuna sarebbe caratterizzata dal fatto che si prevede un precetto, l'obbligo di rendere la dichiarazione entro otto giorni e conseguentemente di regolarizzare la propria posizione, sprovvisto di sanzione. L'introduzione di un'ipotesi contravvenzionale, peraltro, risponde alla logica del nostro codice penale, allorquando la violazione di obblighi amministrativi

provvedimento, che è coerente con il sistema del diritto penale del nostro Paese, anche perché, contrariamente, si verrebbe a creare una discriminazione in negativo nei riguardi dei cittadini italiani, i quali, in caso di violazione di precetti amministrativi, verrebbero invece

concerne la sottolineata violazione dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. È stata qui sostenuta l'idea

al potere legislativo dello Stato e agli organi di polizia dello Stato. In realtà, ciò non è assolutamente fondato, non è vero. Alle associazioni non viene attribuito alcun potere di polizia, ma la possibilità, nell'ambito della regolamentazione di secondo livello e del controllo governativo, di sviluppare attività che tendano a corroborare l'attività delle forze dell'ordine.

parità di trattamento di cui all'articolo 3 della Costituzione. La censura appare assolutamente infondata, perché nel nostro Paese esistono diversi livelli

è previsto il controllo e la verifica giurisdizionale, così come prevede la nostra Costituzione. Mi piace inoltre ricordare gli amici dell'opposizione che hanno sbandierato queste violazioni della nostra Costituzione come nel Paese a più lunga vocazione costituzionale, il Regno Unito, il recente *Human Rights Act* preveda restrizioni della libertà personale di gran lunga maggiori rispetto a quelle previste nel nostro Paese per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico.

introduce il diritto di associazione e di espressione del pensiero e della libertà religiosa), sono previste misure molto stringenti per contrastare i fenomeni di immigrazione clandestina che determinano fenomeni di devianza ed un aumento della criminalità. Non vorrei qui ripetere, lo ho già fatto in altri interventi, che se la popolazione carceraria nel nostro Paese è arrivata a 62.000 unità ciò è dovuto soprattutto a fenomeni di devianza connessi all'immigrazione clandestina. Noi con questo provvedimento diamo corpo a dei princìpi fondamentali, come dicevo all'inizio del mio intervento, che garantiscono, accanto ai diritti di libertà, il diritto alla sicurezza dei cittadini. Non c'è compressione dei diritti fondamentali perché c'è la garanzia della tutela e del controllo giurisdizionale su questi atti; non c'è violazione del principio

i senatori del Gruppo del Partito Democratico voteranno convintamente a favore delle questioni pregiudiziali presentate da tutti i Gruppi delle opposizioni al disegno di legge che stiamo esaminando. I colleghi intervenuti hanno motivato con ricchezza di elementi e fondatezza di analisi le ragioni per cui occorre non procedere all'esame ulteriore del testo. Voglio ricordare brevemente alcune delle ragioni poste a sostegno delle nostre pregiudiziali. In primo luogo, l'introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale, la procedura particolare ed eccezionale prevista, è da un canto inefficace e dall'altro in contrasto con il principio di eguaglianza previsto dalla nostra Costituzione. Ciò, inoltre, può incidere gravemente sull'esercizio di diritti fondamentali, come il diritto alla salute. Le considerazioni svolte dai colleghi della maggioranza non ci portano a modificare la nostra idea. luogo, il prolungamento oltre ogni ragionevole durata della procedura di identificazione e di espulsione nei centri appositamente realizzati trasforma l'esigenza di limitare la libertà di un cittadino per il tempo strettamente necessario in una vera e propria detenzione amministrativa, non dipendente dal comportamento di cui il soggetto interessato è responsabile. l'istituzione delle cosiddette ronde è in palese e insuperabile contrasto con il principio che assegna solo ed esclusivamente allo Stato l'uso della forza a tutela dell'incolumità e della sicurezza delle persone e sempre nel rispetto della dignità delle persone Prima ancora che norma costituzionale e principio generale dell'ordinamento, tale monopolio è tratto distintivo degli stessi fondamenti della nostra civiltà giuridica. Il complesso delle norme che così sinteticamente ho richiamato, signor Presidente, è riuscito in un piccolo straordinario miracolo: contro di esse si è levata la voce unanime di tutte le opposizioni parlamentari. Dubbi e contrarietà sono state espresse anche da parte di colleghi dei Gruppi di maggioranza, che nell'altra Camera e nelle votazioni a scrutinio segreto hanno più volte manifestato evidente contrarietà e solo con il voto di fiducia sono stati ricondotti alla disciplina.

Contro tali norme si è inoltre levata la voce unanime di tutte le organizzazioni degli appartenenti alle forze di polizia. In più occasioni, in convegni, in incontri persino, onorevoli colleghi, in manifestazioni di piazza, i sindacati degli appartenenti alle forze di polizia, da Torino a Catania, hanno manifestato preoccupazione, sconcerto e indignazione. Questo Governo e questa maggioranza da un lato operano un taglio senza precedenti alle risorse destinate al comparto della pubblica sicurezza e dall'altro fanno regali pericolosi alla demagogia, consentendo che si propaghi l'idea di una giustizia fai da te, tanto cara a quell'ideologia predemocratica, da *far west*, che riecheggia in alcune forze politiche. Contro di esse si è levata la voce unanime di tutte le organizzazioni internazionali, dall'Unione europea alle Agenzie dell'ONU, che spesso, non con il linguaggio felpato della diplomazia,

onorevoli colleghi, si è levata la voce di tutte le organizzazioni umanitarie e di tutte le fedi religiose, da quella degli appartenenti alle Chiese protestanti - una per tutte la Tavola Valdese a quella della Chiesa cattolica, che a più riprese e con interventi anche della massima autorevolezza ha richiamato al rispetto della persona umana. Un bel capolavoro, onorevoli colleghi, non c'è che dire. c'è che dire. Per tali ragioni, noi voteremo a favore delle questioni pregiudiziali che sono state presentate, per dare fiato anche in quest'Aula alla stragrande maggioranza del Paese che del Paese che ragiona, ad un Paese che vuole e richiama più attenzione sulla domanda di sicurezza, che chiede e reclama dal Governo e dal Parlamento comportamenti coerenti, severità e rigore, sempre e contro chiunque, ma chiede di agire nel rispetto della dignità umana e dei valori fondamentali della nostra democrazia. Noi voteremo a favore delle questioni pregiudiziali perché l'impianto complessivo della vostra politica di sicurezza si sta rivelando clamorosamente sbagliato ed in contrasto con quella diffusa domanda di sicurezza sulla quale avete chiesto il voto agli italiani e che oggi state tradendo. Sull'immigrazione scegliete la strada del reato, il cui solo effetto annuncio avrebbe dovuto avere ripercussioni mirabolanti e vi trovate con un numero di ingressi clandestini che non si registrava in Italia da molti anni. Quando finalmente scegliete la strada degli accordi e della cooperazione i risultati, al contrario, arrivano. Anziché avviare una seria riforma dell'ordinamento della pubblica sicurezza che organizzi in modo più moderno ed efficace le forze di polizia e che, a parità di risorse, migliori la distribuzione sul territorio, innalzi la capacità preventiva e renda più professionali e meglio equipaggiati ed addestrati le donne e gli uomini dei nostri corpi di polizia, scegliete lo *slogan* e lo *spot* delle ronde e dei muscoli. Questo disegno di legge, questa idea della sicurezza noi oggi li vogliamo fermare anche con il nostro voto.

Presidente, onorevoli senatori, questo disegno di legge, al quale il Governo, com'è noto, attribuisce grande importanza, è stato il primo ad essere approvato nel primo Consiglio dei ministri che si tenne nel maggio dell'anno scorso a Napoli nell'ambito di un più ampio pacchetto di norme in materia di sicurezza. Tutte quelle norme sono entrate definitivamente in vigore nel nostro ordinamento e hanno dato buona prova nel contrasto alla criminalità

componenti, nel febbraio di quest'anno. La Camera dei deputati ha approvato poche e limitate modifiche al testo licenziato dal Senato pertanto il Governo ritiene opportuno, a questo punto, giungere alla definitiva approvazione del testo in tempi rapidi, per consentire che le norme alle quali ho fatto riferimento possano assumere definitiva efficacia nell'azione comune di contrasto alla criminalità.

apre una nuova finestra"). La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 9 luglio. È stato innanzitutto organizzato il dibattito sulle tre questioni di fiducia poste dal Governo sui tre articoli di cui si compone il disegno di legge in materia di sicurezza pubblica. La discussione generale inizierà immediatamente con prosieguo della seduta fino alle ore 14, sospensione dalle ore 14 alle ore 15 e quindi ripresa della seduta fino alle ore 16, orario entro il quale si concluderà la discussione medesima. Alle ore 16 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti renderà una informativa sul tragico incidente di Viareggio. Successivamente potranno intervenire i rappresentanti dei Gruppi per cinque minuti ciascuno. A conclusione di tale dibattito, previa breve sospensione della seduta, si svolgerà - presumibilmente intorno alle ore 17,15 - la prima chiama sulla fiducia relativa all'articolo 1 del disegno di legge. Proclamato il risultato, si svolgerà la seconda chiama sull'articolo 2. La seduta sarà quindi tolta. La terza chiama sull'articolo 3 avrà luogo domani mattina in apertura di seduta, a partire dalle ore 9.30. Alla proclamazione del risultato la seduta sarà sospesa e riprenderà alle ore 12 per le dichiarazioni di voto finali con trasmissione diretta televisiva. Le mozioni in materia di difesa, già previste dal calendario della settimana corrente, saranno discusse nella seduta pomeridiana di martedì 7 luglio. Il calendario della prossima settimana prevede inoltre la discussione - ove approvati e trasmessi in tempo utile dalla Camera dei deputati - del disegno di legge collegato in materia di internazionalizzazione di imprese ed energia

relativo alle interrogazioni alle quali è stata data risposta dal Governo, lamentando il fatto che a quel momento, su dieci interrogazioni presentate nell'arco dell'anno, non una aveva avuto risposta.

avvertendo che, a seguito dell'intervento del Presidente, sulle dieci interrogazioni che attendono da mesi una risposta ho avuto una sola risposta da parte del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Credo che in questo modo la funzione del sindacato ispettivo venga sostanzialmente azzerata e questo non mi sembra un esito accettabile da parte nostra.

discusso, prima in Commissione, poi in Aula, per cui verosimilmente si tratterebbe dell'inutile e frammentaria ricostruzione di un percorso già largamente noto. La sicurezza è un qualcosa che va al di là anche di quello che oggi siamo chiamati specificamente ad esaminare. È un aspetto che il Governo e la maggioranza hanno pienamente colto nel momento stesso in cui hanno affrontato nella sua globalità il problema di una società più sicura. Una società più sicura è una società nella quale la giustizia funziona meglio

in cui il risparmio è garantito: e anche in quella direzione siamo già andati, dimostrando una tenuta migliore rispetto ad economie più forti delle nostre. Ed è una società nella quale

Ma venendo al provvedimento che oggi siamo chiamati definitivamente ad esaminare e votare, esprimendo fiducia al testo che il Governo ci sottopone, direi che il filo ricostruttivo che sostanzialmente ne costituisce l'ossatura portante è costituito È costituito, intanto, da un'analisi lucida, quasi fotografica, delle principali questioni nelle quali poi la domanda di sicurezza si è andata drammaticamente articolando e alle quali non possiamo più tardare a dare una definitiva risposta andando in quella direzione che il Paese tutto ci chiede. ci chiede. La prima delle questioni che dovevamo affrontare in modo assolutamente onesto dal punto di vista intellettuale era allora il nesso inscindibile che intercorre tra due fenomeni: quello della criminalità diffusa (saldata anche, e sempre più frequentemente, alla criminalità organizzata ormai non più soltanto nazionale ma transfrontaliera), radicata nel nostro Paese, e i fenomeni legati all'immigrazione clandestina, dato del quale siamo tutti pienamente consapevoli. Lo abbiamo fatto affrontando il fenomeno in sé e per sé, perché giustamente questa mattina in quest'Aula un collega ha ricordato che vi è un disvalore preciso e un'offensività evidente nella condotta di chi, comunque, varca illegalmente le frontiere di questo Paese e illegalmente in questo Paese soggiorna. Questo era il primo presupposto che dovevamo porci, perché non c'è nessuna comunità, nemmeno in quella più tollerante ed aperta - sicuramente la nostra lo è, perché noi siamo figli e nipoti di migranti e sappiamo quanto sia importante la cultura dell'accoglienza - che possa accogliere tutti indiscriminatamente, garantendo condizioni dignitose di vita e di lavoro. Questo, ahimè, l'immigrazione clandestina non lo consente. Le leggi di questo Paese debbono necessariamente essere rispettate da tutti, anche e soprattutto da coloro che a questo Paese guardano come a una soluzione per risolvere quei drammatici problemi che nei loro Paesi d'origine, purtroppo, gravemente permangono. Sarà una misura efficace e deterrente quella penale di natura contravvenzionale che abbiamo introdotto? Sarà il tempo a dircelo ma, intanto, è una prima concreta risposta che andiamo a dare e che si coniuga, peraltro, a tutta una serie di altre norme che vanno a meglio monitorare, da un lato, e a determinare nelle sue articolazioni, dall'altro, la permanenza e il soggiorno degli stranieri in Italia, a tutela prima non solo e soltanto dei cittadini italiani ma anche di tutti quegli immigrati che legalmente vivono nel nostro Paese e che sappiamo essere una grande risorsa per l'Italia tutta. A questo aspetto, a questa prima fotografia dello stato dell'arte, ne abbiamo aggiunto un'altra, che risponde ad una delle altre articolazioni drammatiche di quella domanda drammatica di sicurezza, vale a dire la tutela più forte dei soggetti più deboli in tutte le loro estrinsecazioni di vita quotidiana (come i minori e gli anziani). In quella direzione noi siamo andati con fermezza ma, soprattutto, con concretezza (che è l'aspetto fondamentale che caratterizza la filosofia di impianto di questo provvedimento). di questa seconda fotografia, in questa sorta di album che voleva in qualche modo rappresentare il problema della sicurezza nel nostro Paese, ne abbiamo affrontato un altro,

introdotto quello per noi rappresenta uno dei portati essenziali dell'essere in politica, vale a dire la cultura della partecipazione e dell'impegno, nella misura stessa in cui abbiamo sanzionato, attraverso l'impossibilità di partecipare poi ad appalti pubblici, coloro che la criminalità organizzata non denunciano. La cultura della partecipazione, come ripeterò conclusivamente, è la strada da seguire, perché si contrappone alla cultura dell'omertà. Sempre in questo ideale album fotografico, ci siamo resi conto quanto, nel contesto di una società sicura, che non è soltanto quella che protegge dai fatti più gravi, sia importante porre fine, una volta per tutte, a quei fenomeni di vandalismo quotidiano che deturpano le nostre città e al tempo stesso le rendono invivibili, coniugando questo percorso a quello di contrasto a quella criminalità diffusa che troppo spesso, riduttivamente ed erroneamente, viene definita microcriminalità, ma che tale non è, inasprendo la normativa in materia di furti e rapine. Dobbiamo infatti essere consapevoli che per una anziana pensionata il furto apparentemente insignificante, proprio da due righe di cronaca nera, della sua borsetta con la pensione rappresenta un evento di una lesività assoluta

Siamo andati ad affrontare anche un altro aspetto drammatico, che purtroppo da anni caratterizza la vita del nostro Paese: quello legato al costo altissimo della sinistrosità in materia stradale, che fa pagare un prezzo spaventoso sotto ogni profilo, prima di tutti quello affettivo come tributo di sangue, di morte e di sofferenze, e poi quello economico. Anche su questo aspetto siamo andati ad incidere non a parole, ma con i fatti.

il pensiero e l'ideazione, come ho detto, è quella della partecipazione dei cittadini, il senso di appartenenza alla comunità, la cultura dell'impegno e dell'assunzione di responsabilità che si contrappone a quella del disimpegno, dell'indifferenza e spesso, purtroppo, dell'omertà. Questa cultura della partecipazione, dell'impegno e dell'assunzione di responsabilità rappresenta una stella polare del nostro cammino in politica, ed è per questo che convintamente voteremo Grazie,

dibattuti provvedimenti degli ultimi anni, di cui credo che dentro e fuori il Parlamento tutti conoscano tutto, almeno per quanto attiene agli aspetti più mediatici

al successo conseguito dalla Lega Nord in prima battuta nella tornata elettorale del 6 e 7 giugno scorsi. Senza nulla togliere alle alte funzioni di quest'Aula, potremmo legittimamente asserire che le norme all'ordine del giorno, bandiera elettorale del nostro movimento e della coalizione vincente, sono reduci dalla più esplicita ed inequivocabile ratifica popolare. Al tempo stesso, e specularmente, sarebbe sensato convenire sul fatto che l'ostinarsi della sinistra nel rincorrere atteggiamenti di gratuita ostilità verso misure necessarie e largamente auspicate costituisca niente più di una maldestra perseveranza in quell'errore, pesantemente stigmatizzato dal giudizio dei cittadini. Anche in questa circostanza, imperterrita, l'opposizione trascina la propria carretta di assortite sentenze di discriminazione, accuse di squadrismi e anatemi di xenofobia. Questa è probabilmente la sola paccottiglia, prodotto di contraffazione, che non riesce a trovare mercato. Che dire a chi attribuisce alla maggioranza la volontà di criminalizzare lo straniero in quanto tale? Certo, introduciamo il reato di immigrazione clandestina, adeguandoci finalmente ai Paesi civili, ai diversi Paesi europei. Nel bel Paese no: doveva rimanere la terra di nessuno, dove chiunque entra a piacimento maturando la convinzione che qui sia lecito fare il comodo proprio. Nella logica distorta di questo modo di pensare della sinistra pare sia il medico a causare la malattia, l'insegnante a generare l'ignoranza, lo spazzino a produrre sporcizia. Stabilendo il delitto di immigrazione clandestina l'irregolare diventa un delinquente. Protesta infatti l'opposizione! Dove l'occhio vede, il cuore duole. Ferrea logica. Altrettanto inoppugnabile un dato che non viene mai considerato dai detrattori del disegno di legge n. 733-B, anche se trattiamo pur sempre del rapporto tra immigrazione e delinquenza.

Con questo, colleghi dell'opposizione, evito ogni altra polemica sulla presunta equazione clandestini-criminali. D'altro canto reputo profondamente scorretto il tentativo di rappresentare in maniera riduttiva, oltre che distorta, l'effettiva portata di questo provvedimento, circoscrivendone il confronto politico e le stesse pretestuose critiche al mero ambito del contrasto all'immigrazione clandestina. Non è solo questo. Tale emergenza esiste e viene adeguatamente affrontata, ma l'azione in questo campo non costituisce solo l'aspetto qualificante di questo disegno di legge sicurezza, e sorprende come un'informazione tanto solerte nel procreare mediatiche figure di eroi antimafia abbia riservato il ruolo della comparsa alle risolutive misure che il pacchetto sicurezza mette in campo contro la grande criminalità organizzata. Distrazione ancora più inqualificabile in considerazione delle gravi minacce ricevute pochi giorni addietro dal Ministro della giustizia e dal suo vice capo di gabinetto, cui va l'espressione della nostra partecipe solidarietà; minacce motivate precisamente dalle severe restrizioni che questo provvedimento dispone nei confronti dei mafiosi detenuti. All'annosa questione della capacità dei boss di conservare e gestire il controllo criminale dall'interno delle carceri ora lo Stato offre una una risposta con un bel giro di vite che questo disegno di legge n. 733-B esercita sullo stesso carcere duro, sanando le smagliature evidenziate nel regime di 41-*bis*, e così via, come abbiamo già ampiamente riferito in Aula. in Aula. Mentre lo Stato si accinge a giocare con questo disegno di legge una partita decisiva contro la mafia, lo stesso provvedimento viene fatto segno di spaventose bordate. Attacchi naturalmente condotti al riparo di improbabili motivazioni umanitarie relative a pretesi diritti dei clandestini. Lo stesso Ministro dell'interno ha tenuto a sottolineare l'importanza delle norme antimafia contenute nel pacchetto, concordate con il procuratore nazionale Piero Grasso, con le associazioni antiracket ed ha ammonito sostenendo che chi avversa questa normativa è più dalla parte dei mafiosi che da quella dei cittadini onesti. Credo che andrebbe ascoltato con molta attenzione quel Ministro che, umile e perseverante con i suoi collaboratori, ha conseguito risultati senza precedenti dal dopoguerra ad oggi. Due dati da soli pesano ben più del profluvio di parole pronunciate e scritte sulla lotta alla piovra. Si tratta di beni per 4,5 miliardi di euro sequestrati ai boss e di oltre 170 pericolosi pericolosi latitanti catturati. Tutto ciò ed altro ancora in appena un anno. Il disegno di legge in discussione si presenta con questo biglietto da visita, che ne qualifica lo spirito e gli obiettivi. Teniamone conto, colleghi senatori, anche se comprendo che ad alcuni apparirà irrinunciabile la golosa polemica intorno a temi più idonei a speculazioni fantasiose. Non difetta, per quanto ne dica l'opposizione, neppure la volontà di persistere, con normativa mirata, nella prevenzione dell'odioso fenomeno della violenza sulle donne. Potremmo tuttavia rilevare che il freno all'immigrazione clandestina, di per sé, opererà apprezzabili effetti in questo senso, considerato che dai dati ISTAT risulta come il 40 per cento delle violenze carnali consumate sull'intero territorio italiano sia compiuto da immigrati, appena il 6 per cento della popolazione residente. In città come Milano e Roma la percentuale degli stupri compiuti da stranieri supera persino quella dei medesimi delitti commessi da italiani. In conclusione, credo che prima di esprimere sentenze viziate da pregiudizio e demagogia su questo provvedimento sarebbe opportuno riflettere sul giudizio che i cittadini, stanchi di restare in balia della criminalità e dell'invasione straniera, hanno riservato a questa sinistra, voltandole le spalle.

Nel complesso, l'impianto ha visto prevalere la politica degli annunci roboanti, della bandiera elettorale, come l'ha definita chi mi ha preceduto, e delle e delle promesse aleatorie, perdendo ogni efficacia sul piano della concretezza, il che rappresenta un paradosso. All'atto pratico il Governo ha dimostrato di essere estremamente lontano dall'ideale del pragmatismo e dell'efficienza che quotidianamente si sforza di trasmettere al Paese ed ha dimostrato quanto sia difficile tradurre gli slogan elettorali, la bandiera elettorale, in norme coerenti ed applicabili alla nostra realtà. Basti pensare alla norma (tralascio il tema delle ronde, ampiamente trattato, perché mi sembrerebbe di sprecare tempo) che introduce in Italia il cosiddetto reato di clandestinità. Al di là delle valutazioni morali (il collega Mazzatorta sa quanta stima ho per lui) ci sono due modi per affrontare il problema: quello etico

Ha mai pensato chi ha ideato questa norma che le nostre carceri sono sovraffollate e che in questo momento contengono 60.000 detenuti quando ne possono contenere solo 45.000? Ha mai pensato che potremmo andare incontro a rivolte nelle carceri? Grandi e gravi incoerenze presenta anche la norma che allunga a sei mesi il periodo di permanenza nei centri di identificazione.

più pigro, meno vicino al nostro Paese, ne subirà le conseguenze. Allora bisogna pensare a trattati con gli Stati stranieri perché ci sia una collaborazione reale ed effettiva. Ciò che mi turba è il pensiero che l'introduzione del reato di immigrazione potrà comportare problemi seri soprattutto negli apparati sociali: penso ai presidi o ai medici. Come si può ritenere che un medico non denunzi un reato? Come si può prevedere che rischi di incorrere in una omissione in atti d'ufficio?

Questa è miopia, ovvero è una bandiera elettorale che nulla ha a che vedere con la concretezza. Mi sarebbe piaciuto, onorevoli colleghi, che su tali questioni e su altre, per le quali non c'è tempo di discutere, avessimo potuto affrontare insieme i problemi, che ne avessimo potuto discutere come si fa in un Paese normale, per assicurare all'Italia, insieme, un futuro sicuro.

ancora una volta, al confronto si è preferito un atto di prepotenza, al dialogo si è preferita l'imposizione di una legge che presenta chiari elementi di immoralità e certamente elementi di incostituzionalità. È una legge

siano temi che non debbano avere una coloritura politica. Quelli della riduzione e della prevenzione dei fenomeni di illegalità sono temi che dovrebbero essere all'ordine del giorno delle politiche di qualsiasi Governo, di centrodestra o di centrosinistra, e di qualsiasi forza politica. L'Italia dei Valori, credo sia noto, è particolarmente sensibile ai temi della sicurezza e della legalità. Ci siamo da sempre impegnati su questi argomenti con proposte politiche legislative degne di nota. Però abbiamo la sensazione, in questo momento, di vivere in un incubo; lo dico molto serenamente e credo che molti cittadini stiano vivendo la nostra stessa sensazione. Ci sentiamo spettatori

Le ronde non le ha certo inventate la Lega Nord, ma possiamo dire che le ha proposte decisamente fuori tempo ed è questo che ci spaventa.

Sottosegretario - di periodi in cui non esisteva lo Stato di diritto, non esisteva un sistema democratico, non esisteva una Carta costituzionale che individuasse con precisione chi doveva garantire l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

istituì un regime di ferrea disciplina tra i suoi liceali per dimostrare come fosse potuto accadere che un intero Paese avesse obbedito ciecamente a Hitler. fece di essi un gruppo militarizzato e in pochi giorni constatò con sgomento che l'obbedienza cieca galvanizzava i ragazzi, innescando derive pericolose e forme di violenza, e ovviamente sospese l'esperimento. Questo è un film, ma è anche una storia vera. Il pericolo che noi vediamo vera. Il pericolo che noi vediamo insito nella costituzione delle ronde è proprio quello che il film ci racconta:

in linea generale su tutto il provvedimento, sia assolutamente contraria in particolare su questa parte. I nostri emendamenti, che purtroppo non avremo l'occasione di discutere perché è stata posta la fiducia, andavano proprio in questa direzione. le ronde nascano da una concezione distorta della sicurezza, quale bene privato per la cui difesa diventa possibile mettere addirittura in discussione quel carattere dello Stato che lo differenzia da ogni altro ente, cioè il monopolio della forza, con tutto ciò che ne consegue in termini di arbitrarie limitazioni della libertà personale dei cittadini, di persecuzione di comportamenti semplicemente non ortodossi, ma soprattutto di sicura costituzione di ronde politicizzate.

quale risulta che sono state presentate le ronde della Guardia nazionale italiana, già ribattezzate ronde nere, un'associazione di cittadini vicina al Movimento Sociale Italiano-Destra Italiana.

ronde proposte nel provvedimento di cui stiamo discutendo saranno una deriva verso la violazione dell'articolo 18 della Costituzione.

simile norma, circa la natura stessa della libertà di associazione, il significato dei suoi limiti costituzionali e la necessità di bilanciarne l'esercizio con gli altri diritti inviolabili, *in* *primis* la tutela della libertà personale. mancanza di consapevolezza ci appare ancora più evidente se ricordiamo una decisione del Parlamento europeo piuttosto recente (del 2007), adottata in relazione al procedimento penale che alcuni parlamentari della Lega Nord avevano subito per la nota vicenda delle camicie verdi. - cito testualmente - «la partecipazione a un movimento i cui membri indossavano un'uniforme di stile militare e che a quanto pare intendeva raggiungere i propri obiettivi mediante l'uso potenziale potenziale o effettivo della forza è chiaramente in contraddizione e incompatibile con il ruolo e la responsabilità inerenti a un mandato parlamentare pertanto non si può ritenere che tale partecipazione costituisca legittimo esercizio del diritto di libertà di espressione, né normale esercizio delle funzioni di un deputato eletto in un Parlamento che rappresenta i cittadini».

una sollecitazione manifestata dal CSM sulla mancanza in questa norma di qualsiasi requisito negativo preclusivo alla partecipazione a simili associazioni. In buona sostanza, anche un soggetto condannato per violenza può partecipare a queste ronde di cittadini. Voi capite che è una pazzia. modo, qualunque cittadino, senza alcun tipo di esperienza, senza alcuna cultura giuridica, senza nulla di nulla, può partecipare a tali associazioni.

esperienza e con una formazione culturale di un certo tipo; niente di tutto ciò è contenuto nella norma. norma. Le ronde nascono - crediamo - da un atteggiamento di una classe politica, la maggioranza di centrodestra, che è inconsapevole degli esiti di disgregazione a cui può condurre il disinteresse per il rispetto della legalità costituzionale. L'Italia dei Valori è presente in quest'Aula e nell'altro ramo del Parlamento per tutelare il rispetto della legalità costituzionale e svolgerà il suo ruolo fino in fondo. *(PD)*. Signor Presidente, colleghi senatori, per quanto ormai il rosario costituito dalla richiesta di voti di fiducia da parte della maggioranza nei confronti del Parlamento si sia allungato, credo che in questa occasione sia necessario un supplemento di riflessione.

accessorie; stiamo trattando della stessa natura che caratterizzerà la nostra futura azione politica. Siamo di fronte a un grande imbroglio, imbroglio, che un Governo incapace di gestire la propria maggioranza sta rifilando agli italiani: da una parte, alimenta l'insicurezza con la criminalizzazione degli immigrati, con la schedatura dei senza tetto, con la creazione di fatto di un clima di tipo emergenziale; dall'altra, rendendosi eccellente dal punto di vista della schizofrenia, impoverisce il comparto difesa e sicurezza, toglie risorse alla polizia, crea le cosiddette ronde, sulle quali tornerò - ed infine - non perché meno importante - propone al Paese una legge sulle intercettazioni, che si articola con l'individuazione di un complicato ma efficace sistema per impedire che la sicurezza del nostro Paese possa essere garantita agli italiani.

la desertificazione dell'Aula che normalmente si crea, ma soprattutto la spoliazione, l'espropriazione che questa maggioranza determina continuamente nei confronti del Parlamento renderebbe il Parlamento medesimo nullo. Io non lo penso e siccome ritengo che un *redde rationem* ci sarà ci sarà e che ad un certo punto le coscienze di tutti verranno chiamate a rispondere di ciò che hanno fatto, siccome penso e spero che quel *redde rationem* possa svilupparsi in maniera democratica, serena e tranquilla e non violenta come altre volte la nostra storia ci ha mostrato, credo che quando verrà il *redde rationem* i parlamentari della cosiddetta maggioranza dovranno rispondere per il razzismo, per la faziosità, per l'indisponibilità all'accoglienza, per un atteggiamento assolutamente opposto rispetto a quello che è previsto nella Costituzione. Si può passare inosservati in un'Aula del Parlamento, si può essere dileggiati o con la smorfia o con il silenzio, ma le parole restano. Questa, signor Presidente, cari colleghi, è una legge vergogna! È una legge che disarticola, che polverizza l'impalcatura e l'architettura del nostro Stato. È una legge che dissolve la storia dell'accoglienza del nostro Paese. Paese. E sarebbe singolare, se non fosse triste e tragico, vedere che dalla stessa parte del Parlamento che appena un paio di mesi fa ci chiamava assassini perché affrontavamo in un certo modo il problema del testamento biologico, oggi venga un atteggiamento chiuso,

quello che penso, e su ciò che penso e su ciò che dichiaro un giorno sarò chiamato a rendere conto, come lo sarete voi, al popolo sovrano. Al popolo sovrano, visto che qualcuno amabilmente mi interrompe. E a quel punto sarà difficile spiegare che il Popolo della Libertà ha dovuto cedere da una parte perché la Lega altrimenti non avrebbe ceduto dall'altra. Tutte queste alchimie, queste forme di insana chimica politica non serviranno di fronte alla coscienza del Paese.

che viceversa è il primo bersaglio di questa azione. Avrei voluto aggiungere qualcos'altro, signor Presidente, ma non intendo metterla nella condizione di togliermi la parola. Spero che le parole che ho detto possano, in qualche modo, costituire se non altro oggetto di riflessione,nei confronti di un Parlamento che della riflessione sembra volerne fare a meno.

che a suo tempo, andando molto indietro con i ricordi, spesso venivamo anche derisi e dileggiati dagli altri partiti perché sembravamo degli extraterrestri che parlavano di fantascienza.

ha acuito il problema della sicurezza nel corso degli anni. E questa mancanza di sicurezza è legata in maniera strettamente proporzionale all'aumento indiscriminato del numero di immigrati clandestini presenti nel nostro territorio. credo sia un dato di fatto inconfutabile. Gli immigrati sono spinti verso il nostro Paese dello stato di povertà dei Paesi di provenienza, attratti spesso e volentieri dai miraggi trasmessi dai canali televisivi satellitari.

del lavoro nero. Le indagini conoscitive della Commissione antimafia ci dicono anche che molto spesso vengono intercettati da compagini malavitose spesso e volentieri di matrice straniera.

perché effettivamente siamo invasi e travolti da un'immigrazione incontrollata che ci ha portati ad una deriva della sicurezza, quella che abbiamo visto e vissuto in questi ultimi anni. Servono inevitabilmente

che mi ha preceduto, la senatrice Bugnano, che prima ha svolto un intervento di 15 minuti parlando dei gruppi di volontariato a controllo e difesa del territorio, che qualcuno in maniera furbesca ha definito ronde. Ho la la presunzione di essere stato uno dei primi sindaci ad aver adottato le ronde, circa tre anni fa, nel proprio territorio e sono contento di averlo fatto. Ogni tanto

Concludendo, bisogna riconoscere che è passato un anno da quando abbiamo iniziato la discussione di questo decreto. Sulla sicurezza tutti abbiamo discusso e sicuramente abbiamo avuto tanto tempo, senatore Serra: un anno credo sia più che sufficiente

il voto di fiducia, che era allora in prima lettura, affermando che sul tema dell'immigrazione l'articolato contiene disposizioni inattuabili, con formulazioni pasticciate ed è condito dal disprezzo dei diritti umani, con un chiaro avvertimento: la vita dell'immigrato sia difficile, la sua cacciata facile. Potrei riprendere quell'intervento punto per punto, ribadendo le ragioni - incessantemente ripetute dalla nostra parte politica - di una netta e ferma opposizione a questa legge: la pericolosa criminalizzazione dell'irregolarità, nella quale si può cadere anche per semplici inosservanze amministrative, e l'impraticabilità della norma, qualora davvero la si voglia applicare; la minacciosa istituzione delle ronde; l'insensato ed impraticabile registro dei senza fissa dimora; la tassa su concessioni e rinnovi dei permessi di soggiorno; le ulteriori difficoltà frapposte al conseguimento del titolo di lungo soggiornante; la connessione - fatale per il sistema statistico nazionale - tra iscrizione anagrafica e idoneità sanitaria dell'abitazione; la trovata del permesso di soggiorno a punti, di cui nemmeno i proponenti sanno bene cosa fare. E alle disposizioni vessatorie o inique contenute in questa legge fanno da contorno altre norme, contenute in altri involucri del pacchetto sicurezza, tra le quali spicca l'iniqua ed anticostituzionale aggravante di pena per gli irregolari che commettono determinati reati. Altri, assai meglio di me, analizzano e analizzeranno le contraddizioni e le inadeguatezze giuridiche di questa legge; pertanto nel tempo che mi resta svolgerò un ragionamento diverso. Per farlo, mi è stato utile entrare nella *privacy* dei componenti di questo Senato, per cui mi scuso con tutti voi, colleghi, per questa intrusione. L'ho fatto, però, sulla base di informazioni rese pubbliche e accessibili Ebbene, le senatrici ed i senatori, che mediamente sono nati negli anni '50 e hanno perlopiù completato il loro ciclo riproduttivo, hanno messo al mondo pochi figli: in media, si tratta di 140 figli ogni 100 colleghi che siedono su questi scranni. Questo numero è basato su un campione, ma mi ripropongo in futuro di fornirvi un dato esatto, fondato su una rassegna completa. Ognuno sa che per fare conto pari, da una generazione all'altra, questi figli dovrebbero essere almeno 200 ogni 100 titolari del laticlavio senatoriale, due a testa (uno per chi è titolare del laticlavio e uno per il o la partner). Nonostante i lodevoli sforzi di qualche collega, qualcuno dei quali siede tra i banchi della mia parte politica, i senatori sono di un terzo al di sotto del *plafond* ideale. Questo lato oscuro della nostra produzione senatoriale - non quella legislativa naturalmente, che è ottima e abbondante - ha un elemento di consolazione: noi, democraticamente eletti, siamo un fedele campione degli italiani, dei quali replichiamo esattamente il comportamento demografico. Si tratta di quello stesso comportamento riproduttivo parsimonioso che farebbe sì che nel prossimo quindicennio, qualora le porte restassero ermeticamente chiuse all'immigrazione, come alcuni della maggioranza auspicano, i già scarsi giovani di questo Paese diminuirebbero mediamente ogni anno di 150.000 unità. È più o meno come se in un anno sparisse l'intera popolazione di Reggio Emilia, quello successivo quella di Ravenna e poi quelle di Salerno, di Foggia, di Cagliari e poi ancora di Livorno e di Perugia. Non proseguo. Quasi tutti comprendono che un declino di questo genere è insostenibile: entrerebbero in crisi molti settori produttivi, si indebolirebbe l'economia, ne soffrirebbe il *welfare*, rimpicciolirebbe l'Italia rispetto ad altri Paesi, saremmo - ohibò - retrocessi dai G8 ai G20. Fortunatamente, c'è un pilastro di sostegno, che si chiama immigrazione e che tutti noi vogliamo regolare e conforme alla legge, limitando, per quanto possibile, l'irregolarità; quanto possibile, l'irregolarità; magari riformando il canale tortuoso ed impervio dell'accesso legale che spinge famiglie ed imprese ad assumere gli *overstayers* che possono guardare in faccia e conoscere, senza la lotteria della chiamata al buio; magari allungando la validità dei permessi di soggiorno, sveltendo i rinnovi, rendendoli gratuiti anziché onerosi; magari chiudendo la trappola di un'irregolarità dovuta all'inefficienza e all'accanimento burocratico; magari prosciugando l'economia sommersa, potente calamita dell'irregolarità. Armeggiare con gli articoli del codice penale non serve: anzi, è l'arma di chi è impotente a fare una politica delle migrazioni. Vogliamo poi che il pilastro dell'immigrazione sia solido, composto di migranti in regola con la legge (una legge, certo, non inutilmente vessatoria), per i quali venga favorita l'integrazione, a cominciare dalla concessione della cittadinanza a chi nasce in Italia; venga facilitata l'acquisizione della residenza e della carta di lungo residente; non venga resa problematica l'iscrizione in anagrafe, istigando al sotterfugio; non vengano lesinati i diritti sociali; non venga ristretto il diritto alla riunificazione familiare. Voglio ripetere quello che il Presidente della Camera ha più volte sostenuto, da quel sovversivo che è, cioè che sia opportuno concedere loro il voto amministrativo dopo qualche anno di residenza. Gli immigrati non sono una protesi, da gettar via quando non serve più. Tanto più che - come dimostra la persistente bassa natalità - questa protesi dovrà servire a lungo. Siano invece un trapianto che attecchisce e diventi parte della società. Questa legge contribuisce all'erosione ed all'indebolimento del pilastro migratorio; va contro gli interessi del Paese; contribuisce al discredito e all'avvilimento degli immigrati; non risolve il fenomeno dell'irregolarità; fertilizza il terreno della discriminazione; è una rinuncia ad una politica migratoria di largo respiro. Aggiungo pertanto il mio voto contrario convinto a quello del mio Gruppo.

aggiungo alcune notazioni critiche. La prima riguarda il mito della sicurezza. Qui è stato messo in discussione un provvedimento con l'intenzione, proclamata e retorica, di garantire la sicurezza. Eppure, nello stesso momento, il Senato affronterà tra breve un provvedimento sulle intercettazioni che rappresenta un palese attentato alla sicurezza. Non mi dilungo su questo argomento perché ci sarà tempo per discuterne ma devo ricordarlo perché, nello stesso momento in cui si priva la magistratura e la polizia degli strumenti fondamentali iniziali di apertura per indagare sul crimine organizzato e sulla grandi organizzazioni criminali quali mafia e camorra, non si può dare ad intendere al popolo italiano che si sta lavorando per la sicurezza. Il secondo punto, sempre in termini di criticità della questione sicurezza, riguarda l'identificazione dei fattori dell'insicurezza. È abbastanza curioso che, in una società italiana dove gli elementi della sicurezza sono incrinati in una maniera vasta e profonda in tutto il tessuto sociale, l'identificazione del fattore fondamentale dell'insicurezza venga caricato quasi tutto sulla figura del migrante. Si dimentica che, all'interno del popolo italiano, vi sono formidabili risorse per la criminalità e che noi siamo famosi nel mondo per le grandi organizzazioni criminali, radicate e capaci anche di muovere il mondo politico, oltre che l'economia. Si dimentica che c'è una platea sociale che fa addirittura da tessuto alla base di queste organizzazioni e ci si viene a dire che

drogati in crisi di astinenza o da immigrati, cioè le persone più facili da prendere. Ma che la popolazione carceraria sia così caratterizzata non prova assolutamente niente; prova semmai una cosa diversa, ossia l'iniquità di principio della società italiana, che non riesce a gestire il tema della giustizia in termini giusti. Già chiamare questo disegno di legge «provvedimento sulla sicurezza», quindi, fa parte di un inganno e se lo scorriamo, anche rapsodicamente,

Se il mio collega Livi Bacci, valentissimo professore di demografia, avesse avuto il tempo per parlarne - ne avrà il tempo in futuro, spero - avrebbe potuto spiegare alla platea del Senato che è proprio l'ostacolo al matrimonio e all'iscrizione a scuola che costituisce un fattore di insicurezza. Non ci si può lamentare degli stupri notturni - bisogna poi sapere che in realtà gli stupri li commettono anche gli italiani,

impediamo le misure che potrebbero determinare la coesione sociale dell'immigrato, che entra in un mercato del lavoro difficile, in un mercato del lavoro sommerso, con difficoltà di relazioni. *(Commenti del

di solito prova ad integrarsi in un mercato del lavoro che sembra fatto apposta per metterlo in una condizione di soggezione. Infatti, questo non va dimenticato: è un mercato del lavoro sommerso,

in tutta buona fede, possano immaginare ostacoli al matrimonio degli immigrati. Intanto, ciò rappresenta una negazione del proprio orientamento religioso: non è sulla famiglia che è basata la società? Vengono versati fiumi di retorica al riguardo: viva la famiglia! Quanto è importante la famiglia! impediamo e rendiamo difficile la realizzazione della famiglia e rendiamo difficilissima, tanto per caricare il peso, la realizzazione della riproduzione della famiglia. Che cos'è negare l'accesso a scuola ai bambini figli di clandestini se non negare il diritto alla riproduzione della famiglia? Il prete di Campi Bisenzio parla con i cinesi tramite i loro figli, che vanno a scuola e parlano sia cinese che italiano: non si rivolge ai cinesi adulti. Comunica con le famiglie attraverso i bambini che hanno imparato a scuola a parlare italiano. Quindi, se vi è un provvedimento che si dovrebbe prendere per la sicurezza, non per il bene dell'immigrato, e per la coesione sociale sarebbe proprio quello di fare in modo che gli immigrati possano sposarsi tranquillamente e mandare i figli a scuola.

Questa è la logica con cui si affronta un problema sociale se si pensa che sia drammatico. Se, invece, lo si affronta soltanto con la logica proibizionistica, non dialogante, con la logica dell'opposizione ferma, ferma, siamo di fronte ad un irrigidirsi delle difficoltà. Sulle ronde hanno già parlato i miei colleghi. Ho ascoltato con attenzione la spiegazione mite che ne ha dato l'ultimo esponente della Lega. Sono il primo ad apprezzare

non sempre sarà un momento di dialogo dolciastro, perché la nostra società è difficile, ma la partecipazione deve essere interlocuzione. L'idea di questi bravi cittadini senza macchia e senza paura che occupano il loro tempo libero percorrendo le strade con quella funzione lascia veramente stupefatti. Torno per un momento sul problema degli stupri. Davvero gli immigrati sono gli autori degli stupri? degli stupri? I giovani italiani dei licei e dei ginnasi non esercitano le stesse attività? Nei quartieri metropolitani delle grandi città non ci sono aggressioni di gruppo di italiani a danno di italiane?

Presidente, ciò che a noi preme è che in questo dibattito, che poteva anche essere interessante, vi è stata pochissima onestà intellettuale.

non va bene, non va bene, non va bene, non va bene! Un po' come i vecchi processi al Giro d'Italia, quando c'era Bartali, in cui era tutto da rifare. sono venute osservazioni e cadute di stile anche da personaggi stimabili, da magistrati che riteniamo competenti ed apprezzabili.

Da Genova in poi, elenchiamo tutti i danni che hanno combinato questi ragazzini! Possiamo fare un abbinamento? È poco serio. Penso alla collega dell'Italia dei Valori che è intervenuta

la sinistra è slegata completamente dalla realtà, non ha più un termometro o un sistema di monitoraggio e vede il consenso scemare, dalle politiche alle europee. 26 Province perse dal centrosinistra non significano niente? 9 grossi capoluoghi di provincia persi nelle grandi città e nelle regioni rosse, dall'Umbria alla Toscana, all'Emilia, città come Orvieto, Prato e Sassuolo che cambiano colore significano qualcosa?

e mi sembra che il consenso e le indicazioni politiche siano arrivate. O voi riuscite a cambiare registro ed a essere seri nei ragionamenti e nelle proposte o probabilmente non vi solleverete più.

quale timore si avrebbe nel sottoporlo al voto palese in Aula o anche al voto segreto, visto e considerato che c'è una forte domanda di sicurezza da parte di questi poveri italiani, assediati - Nord, Centro, isole, montagne, mari e pianure - da un'orda di barbari che proviene da tutto il resto del mondo e e che, indipendentemente da ciò che li caratterizza (e, ahinoi, non è soltanto la fame ma anche i conflitti armati), vuole venire nel Paese del Bengodi a stuprare le nostre donne, prenderci il posto di lavoro e, se possibile, a svaligiare tutte le nostre villette o appartamenti in megacomplessi industriali? Questo Parlamento che è con il Presidente del Consiglio probabilmente (silenziosamente o meno silenziosamente) deve aver fatto capire che il "popolo della sicurezza" non è così compatto, che forse ancora

Il popolo a questo punto - c'è stato detto adesso - sceglie chi impone la sicurezza. Posso però ricordare che se proprio si fosse così dediti all'imposizione della sicurezza, magari, quando si è sindaco, si deciderebbe di fare il sindaco piuttosto che il sindaco e anche il senatore, perché nei tre giorni in cui si è assenti dal proprio ufficio al Comune sicuramente può essere messo a ferro e fuoco il paesello dell'ultima valle della Padania. Lo stesso si dica per i vicesindaci della capitale. Questo è un argomento che un giorno bisognerà affrontare, visto e considerato che non si può necessariamente fare bene allo stesso tempo

Questo popolo, ci viene detto, chiede a gran voce misure per la sicurezza perché è sottoposto a minacce di tutti i tipi.

da quando è iniziata la campagna elettorale del 2008 la maggioranza che oggi siede in Parlamento ci ha martellato con la necessità di inasprire qualsiasi pena già esistente e di introdurre addirittura nuove fattispecie di reato. Ricordo che poche settimane fa,

Si registra la sovrappopolazione di una serie di penitenziari che, grazie ai tagli orizzontali, non soltanto non hanno più dotazioni per la manutenzione o l'ordinaria amministrazione,

la bella stagione, con l'aumento degli arrivi (checché se ne dica magnificando i contatti con il compagno Gheddafi) e con l'aumento dello spaccio di sostanze stupefacenti, potrebbe raggiungere i 75.000 ospiti da qui alla fine di agosto. agosto. Vi state candidando a fare dell'Italia - in questo caso, sì - un'ex repubblica sovietica, dove qualsiasi cosa si faccia deve essere punita sempre e solo con una sanzione penale,

le norme alla nostra attenzione risalgono a circa un anno fa. Qualora fossero confortate dal voto favorevole del Senato, esse completerebbero un dispositivo che abbiamo anticipato l'anno scorso e che abbiamo esteso, la scorsa settimana, alle norme del Trattato di Prüm. Si tratta quindi di un pacchetto abbastanza coerente di politiche per la sicurezza. Non mi è facile, nel tempo che ho disposizione, contrastare tutti i gli elementi di immoralità e di incostituzionalità, per dirla con il collega Serra, che l'opposizione attribuisce a questo provvedimento. Devo dire, in parte sulla scia delle considerazioni del senatore Divina, che gran parte degli argomenti utilizzati e gran parte dei sentimenti espressi mi sembrano dettati In particolare, c'è un insistito ed insistente processo alle intenzioni di ronde padane

volontari per la sicurezza dei turisti, come sono stati chiamati dall'assessore alla formazione il quale aveva composto questi corpi di volontari

non mancano, nel nostro Gruppo, sensibilità e valori di umanità che ci portano ad esprimere preoccupazione allo stesso modo del senatore Perduca. Perduca. La Regione Campania, in questa miscela di cinismo e di buonismo, servendosi di fondi destinati a ben altro, ha assunto in servizio

e possono garantire la sicurezza dei turisti. Di fronte a simili manifestazioni, io ho sollecitato alcuni colleghi del centrosinistra a firmare l'interrogazione che ho presentato insieme al presidente Gasparri e ad altri colleghi campani. Contavo molto sul senatore Morando, che mi aveva espresso anch'egli la sua perplessità e la sua indignazione.

con tanta indulgenza e tolleranza allo spregiudicato e cinico clientelismo che è dietro le ronde borboniche, io, che non amo né Borbonia né Padania

La gente le guarda con simpatia, proprio perché magari le preferisce alle ronde padane, che invece non esistono. Non solo:

Allora, con che serietà una collega che molte volte ammiro, la senatrice Bugnano, viene a parlare di privatizzazione, di ritorno al Medioevo, di dissoluzione dello Stato? Stato? Quando si esaminano tali provvedimenti, occorre una certa onestà intellettuale, la stessa con la quale questa mattina un collega che stimo molto, il senatore Mazzatorta, notava come, con scarsissimo rispetto del Senato, tutto il lessico delle pregiudiziali di incostituzionalità fosse, punteggiatura per punteggiatura, targato CSM,

Mi soffermo su questo aspetto. Molte volte le cronache della mia città e della mia Regione - parlo di Napoli e della Campania - si prestano a interpretazioni macchiettistiche, però qui c'è un fallimento della Regione come istituzione, del bassolinismo come restaurazione del Rinascimento, dopo il Medioevo denunciato dalla senatrice Bugnano. La vostra indulgenza è una forma di complicità, perché non potete fare il processo alle intenzioni, ai commi ai commi 40 e 41 e seguenti dell'articolo 3, dopo che avete plaudito a questa cinica regionalizzazione.

molte volte vediamo Regioni che vengono meno ai loro compiti di programmazione e di legislazione e se ne vanno a cercare altri di gestione. Ne deriva un regionalismo di potere e di clientela, che sfrutta cinicamente il buonismo della condizione degli ex detenuti, senza respiro e senza prospettiva. Da questo punto di vista, in materia di priorità della politica della sicurezza, meno che mai tali priorità possono essere indicate dalle Regioni: questa sì sarebbe stata abdicazione dello Stato. Pertanto, non prendo sul serio gli argomenti e i sentimenti sollevati in questo dibattito da parte di chi ha guardato dall'altra parte mentre la Camera legiferava con prudenza e saggezza sull'articolo 3 la Regione Campania si vantava di un cinismo che non onora le Regioni del Mezzogiorno.

non facendo solo una questione di moralità o, peggio, di moralismo. Ho ascoltato il collega Mazzatorta, non oggi ma anche in altre occasioni, quando si riferisce ad un presunto senso di superiorità da parte della sinistra.

Divina), dell'integrazione che esiste in altri partiti di storie diverse, per cui attribuire a una parte il tutto o viceversa spesso non aiuta nel ragionamento, soprattutto qui dove non dobbiamo certamente incendiare i nostri sostenitori, non credo che ci non credo che ci sia questa superiorità nella testa di molti colleghi; se c'è, è sbagliata. Vogliamo ragionare del fatto che siano effettive ed efficaci le norme che vengono prodotte; poi ognuno di noi

potrei sbagliarmi), perché debbo associare la questione dell'immigrazione a quella della sicurezza? I dati sui reati li indicano in diminuzione, salvo l'odioso reato della violenza sessuale, che poi perlopiù in Italia è un problema all'interno delle famiglie,

Tra l'altro, i reati commessi da persone straniere (quindi anche dal facoltoso cittadino abitante a Miami, Stati Uniti d'America, per intenderci, oltre che dai cittadini extracomunitari e comunitari), sono esattamente gli stessi, anzi leggermente meno, in proporzione, di quelli che commettono i cittadini italiani. Tutti abbiamo raccontato delle

tra l'altro con una possibilità di reiterazione dei reati. Allora, se non c'è questa associazione nei fatti, questo è un aspetto semplicemente ideologico e di propaganda. Di per sé non trovo nulla di male nel fatto che una maggioranza proponga tali questioni (tra l'altro questo non a caso è stato il primo decreto-legge, poi cambiato, che è stato proposto al Paese), però poi bisogna fare i conti con l'efficacia di queste norme, cioè se si risolvono i problemi:

consolato per chiedere un documento digitale, per avere una tessera sanitaria che testimoni delle sue vaccinazioni, per risiedere laddove noi diciamo che deve risiedere per sei mesi per poter cercare il suo posto di lavoro. lavoro. Questo eliminerebbe alla radice intanto il mercato degli scafisti e poi permetterebbe i ricongiungimenti familiari che garantiscono contro la malavita o la disperazione, perché chi ha una famiglia delinque di meno (questo vale ovviamente per gli italiani e anche per gli stranieri). Questa è una scelta faticosa, perché significa dare forza al Ministero dell'interno, dargli i denari per poter operare, dare i denari per riformare la struttura dei nostri consolati e delle nostre ambasciate all'estero che cade a pezzi e che non è in grado di garantire nemmeno i nostri cittadini. nostri cittadini. È più faticoso, è un modello alternativo, è un modello che dice: vivaddio, vengono in questo Paese e nel Nord-Est; se riparte la ripresa - la crescita economica che questo Governo vorrebbe dare - avremo la gente che lavorerà,

La verità è che questo modello non reggerà e, con molta sincerità, com'è giusto che sia, quando noi saremo maggioranza cancelleremo una ad una le vostre norme.

lesivo della dignità umana e - quel che è peggio - assolutamente inefficace dal punto di vista della tanto da voi abusata sicurezza dei cittadini. Infatti, istituendo il reato di clandestinità, il disegno di legge promuove una politica di repressione e di intimidazione ed alimenta ulteriormente quel clima di insicurezza e di paura che voi stessi avete creato a fini elettorali e quella xenofobia che purtroppo sempre più spesso compare sulle pagine di cronaca dei nostri giornali. Per di più, il reato di clandestinità, che reato non può essere in quanto si tratta in realtà dello *status* di una persona e non di un comportamento criminale, provocherà un aumento esponenziale dei processi e delle attività giudiziarie, aggravando la situazione già non rosea del nostro sistema giudiziario. Processi che aggraveranno i nostri conti pubblici e ritarderanno le eventuali giuste espulsioni, affiancate da assurde sanzioni pecuniarie che la maggior parte degli immigrati stranieri non potrà permettersi di pagare. Volete solo demagogicamente trasformare il clandestino, spesso un profugo, in criminale e la disperazione in reato. Vorrei ricordare al collega Mazzatorta, per quanto dichiarato stamattina, che soltanto la disperazione spinge gli immigrati a superare illegalmente le nostre frontiere, non ci sono davvero altre motivazioni. la norma veramente scandalosa che state cercando di camuffare in tutti i modi è quella che renderà invisibili migliaia di bambini figli di stranieri, che nasceranno in Italia e non saranno iscritti all'anagrafe diventando di fatto dei fantasmi agli occhi del mondo. Infatti, se l'immigrazione clandestina sarà reato, se per compiere qualsiasi atto di stato civile (non solo per il matrimonio di un cittadino o una cittadina o tra cittadini stranieri) dovrà essere preventivamente esibito il titolo di soggiorno del richiedente, poiché l'articolo 362 del codice penale obbliga gli incaricati di pubblico servizio a denunciare all'autorità giudiziaria i reati di cui hanno avuto notizia dell'esercizio delle loro funzioni, allora sarà impossibile per le madri immigrate non regolari, non solo registrare il figlio all'anagrafe, ma addirittura il riconoscimento, con la conseguenza di perdere la custodia dei loro bimbi che di fatto diverrebbero, secondo le leggi italiane, adottabili. Siamo davanti ad una evidente violazione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, che prevede espressamente l'obbligo di registrazione della nascita di qualsiasi bambino nato in qualsiasi Paese che abbia sottoscritto la Convenzione stessa, a prescindere dalla cittadinanza dei genitori e, ovviamente, dalla regolarità del loro soggiorno. nella Commissione bicamerale per l'infanzia, tutti noi componenti, senatori e deputati d'opposizione e di maggioranza, dopo diverse audizioni degli operatori del settore ed anche del ministro Maroni, abbiamo sottoscritto ed approvato una risoluzione per la tutela dei diritti dei minori stranieri non accompagnati, impegnando tra l'altro il Governo «ad adoperarsi «ad adoperarsi affinché ogni intervento, anche normativo, che influisca sulla condizione dei minori non accompagnati nel nostro Paese, risulti in armonia con i principi della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché con la normativa dell'Unione europea e con le indicazioni del Consiglio d'Europa in materia». Ad oggi, purtroppo, quella risoluzione non ha avuto alcun seguito. Sempre in quell'occasione, nel corso delle audizioni, siamo venuti a conoscenza di dati inquietanti circa l'immigrazione clandestina dei minori e, in particolare, lo stesso Ministro dell'interno ha dichiarato che la scomparsa di una percentuale di minori è ricollegabile ad un possibile traffico internazionale di organi. È chiaro che se non riconosceremo il diritto ad avere un'identità a tutti i minori stranieri in Italia e se l'ordinamento italiano non continuerà a considerare il minore straniero sempre e comunque un minore, ovvero un soggetto che ha la necessità di essere assistito, accudito e tutelato, avremo in Italia bambini senza diritti, senza la possibilità di andare a scuola, che diventeranno facili prede della criminalità organizzata e vittime di abusi e sfruttamento. allora quale utilità possano avere queste norme aberranti dal punto di vista della sicurezza e dell'ordine pubblico. «Non c'è sicurezza senza il rispetto dei diritti umani di ogni persona»: cito il titolo di un documento che tutti abbiamo ricevuto a questo riguardo dalle ACLI di Milano e firmato dall'Azione cattolica ambrosiana, dalla Comunità di Sant'Egidio, dal Movimento dei focolari e dal Gruppo promozione donna. Purtroppo, voi siete sordi a qualsiasi richiamo al buonsenso, a quello del presidente Napolitano come a quello del presidente della Camera Fini, a quello della CEI e del Papa come a quello dell'ONU e dell'Unione europea, e andate avanti senza alcun rispetto per la dignità umana. Se davvero teneste alla sicurezza, dovreste piuttosto mettere in cantiere un pacchetto per l'integrazione e l'intercultura, il vero obiettivo a cui dovrebbe tendere la nostra società, che multietnica e multiculturale lo è già. *(Applausi

è da ieri che sento i senatori dell'opposizione fare lezioni di diritto costituzionale, ma un fatto è certo, cari colleghi: per la prima volta dopo dieci anni, grazie alle buone leggi e all'avveduta azione di Governo, non avvengono più sbarchi di clandestini a Lampedusa. Non ci interessano le vostre critiche: non ci sono mai interessate e non interessano soprattutto al nostro Paese, visto che ormai hanno cancellato le vostre idee. Lampedusa, signori, oggi ha zero immigrati nel CPT e questo risultato porta una sola firma: quella del ministro dell'interno Roberto Maroni, al quale va il ringraziamento mio e del mio popolo.

che solo i fatti ci portano avanti. E questi appunto sono fatti, cari colleghi dell'opposizione; le vostre, invece, sono solo parole. Le scelte del Governo sono quelle giuste. Anche coloro che mostravano scetticismo in merito alla soluzione del problema si sono dovuti ricredere. Solo voi dell'opposizione sembrate rimpiangere la situazione precedente agli interventi del Governo, quella in cui ogni giorno avvenivano nuovi sbarchi nella mia meravigliosa isola; anzi, sembrate quasi voler tornare a quei tempi. Ma noi non lo permetteremo, perché stiamo lottando per fermare questo fenomeno! Voi condannate l'azione del ministro Maroni, ma in nome di che cosa? Quali proposte fate? Quali interventi indicate per risolvere il problema dell'immigrazione clandestina? Ve lo dico io cosa proponete: nulla, come nulla avete fatto in tutti gli anni in cui siete stati al Governo del nostro Paese! «Lampedusa è tornata al nostro Paese come la perla del turismo»: ad affermarlo non sono solo io, che ci vivo, ma è stato il ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi, recentemente in visita sull'isola. Quindi ci sono testimonianze. Le bugie, cari colleghi, hanno le gambe corte: il tempo ci darà ragione. Io sono stata penalizzata nella mia isola, ma oggi mi posso presentare a testa alta. Da oggi l'immagine di Lampedusa può cambiare perché il mar Mediterraneo non presenta più quelle immagini terribili di clandestini e di disperati. Questa è la prova più concreta della grande opera del Governo, ed è inutile diciate che questo fenomeno ricomincerà: sicuramente noi vigileremo. Il nostro Paese si libererà presto. Un plauso va la anche alle forze dell'ordine della mia isola, alla Guardia di finanza, alla Guardia costiera, al comando dei Carabinieri e anche ai Vigili del fuoco di Lampedusa, per il difficilissimo lavoro che svolgono costantemente, anche se non dobbiamo mai abbassare il livello di attenzione. Lo ripeto: non dobbiamo mai abbassare il livello di attenzione. Grazie Grazie all'approvazione di questa legge, una cosa ora è chiara anche ai trafficanti di uomini (perché sapete benissimo che in questi anni voi avete dato forse la possibilità a questi trafficanti di agire indisturbati): il nostro Paese non sarà più un colabrodo, non è più il ventre molle dell'Europa, senza controlli e senza regole sull'immigrazione! Ora, passata l'emergenza, è il momento di ripartire. Bisogna mettere in campo iniziative per promuovere il turismo a Lampedusa, perché la mia piccola isola se lo merita. Ed io lavorerò in tal senso,

Signor Presidente, quello della sicurezza è quasi uno spettro che si aggira, se non per l'Europa, almeno in Italia. Agitato come una clava in campagna elettorale, il problema - reale, virtuale o percepito che dir si voglia - si è tradotto in provvedimenti che vorrebbero scandagliare chissà quali profondità e che, purtroppo, agiscono invece solo sul versante più prossimo all'odierno conformismo. Il tema, infatti, coinvolge non solo e indifferentemente la società nel suo complesso, ricadendo a pioggia sulle fasce più deboli della popolazione che rimangono - occorre sempre dirlo - l'anello più esposto della catena sociale, ma una serie di addentellati che formano insieme il senso stesso di uno Stato di diritto. Voglio dire che non si può affrontare questa questione senza andare a intervenire sull'idea di società che si vuol realizzare e che vi sottostà. Ora, dinanzi alle spinte riformistiche messe insieme e rivendicate dal centrodestra, inverate nella filosofia di Umberto Bossi e della politica dell'"ognuno è padrone in casa sua", francamente mi sfugge il disegno. Soltanto l'altro ieri, sulla prima pagina di quel foglio scapigliato e rivoluzionario qual è il «Corriere della Sera», Piero Ostellino enumerava i ritardi e le colpe di un Paese che si avvia a divenire la brutta copia di una brutta America. Certo, le contraddizioni non mancano: si punta il dito, a ragione, contro l'immigrazione clandestina, ma in comparti come quello agricolo o dell'edilizia, in cui i lavoratori italiani sono ormai un'esigua minoranza, quanti piccoli e medi imprenditori si servono di mano d'opera a nero? Non è questo un tema che attraversa il piano più generale della sicurezza? È notizia di ieri, che si aggiunge al quotidiano bollettino delle morti sul lavoro, quella dei due operai folgorati nel Pavese. Non riguarda in qualche modo la sicurezza? Troppi morti sul lavoro e sulle strade, ma non solo. Caporalato al Meridione, bullismo nelle scuole, carceri sovraffollate, strutture fatiscenti, lentezza dei processi, disagi non solo formali della polizia penitenziaria, ritardi nelle sempre più urgenti riforme di cui abbisognerebbe la disciplina penale per un giusto processo, sostanziale assenza di sanzioni o, comunque, sanzioni inadeguate alla colpa commessa, e via enumerando: non sono questi solo alcuni degli elementi in cui a più vasto raggio può declinarsi il problema della sicurezza che, cacciato dalla porta del provvedimento di legge, inevitabilmente rientrerà dalla finestra della cronaca e dei telegiornali? Mi limito ai proclami di Alemanno e della sua Giunta: non mi sembra che per quantità o qualità i crimini nella capitale siano diminuiti: ciò che è mutata è la risonanza mediatica, trasformatasi da propaganda in minaccia. Per questo riflettevo sul disegno della società che si vuole realizzare, a fronte di una materia così delicata e complessa: non voglio per questo mescolare le carte per appoggiare indirettamente forme di inadeguato garantismo, che si rivelerebbero miopi e soprattutto inefficaci rispetto alla grande trasformazione in atto nella società. E tuttavia promuovere le ronde di cittadini, con le automobili della polizia senza benzina nei garage, è grave non tanto ovviamente per la cosa in sé, ma perché veicola palesemente un'impotenza cui lo Stato non riesce a far fronte: un'impotenza velata dei pericoli che comportano (in una sorta di medioevo prossimo venturo, come si intitolava un libro di Roberto Vacca di qualche anno fa) le forme di faida, il diritto di farsi giustizia da soli, e dunque il pericolo di una giustizia comunque sommaria. Tutti elementi che, in una parola, alimentano sfiducia nelle istituzioni. Una polizza assicurativa non impedisce il verificarsi di sinistri; e comunque il problema della sicurezza non si può risolvere con il semplice - se pur indubbiamente necessario - aumento delle forze dell'ordine sul territorio, né tanto meno con la positiva introduzione del poliziotto di quartiere. Il punto è quale natura deve assumere, quale identità vogliamo che assumano quel territorio e quel quartiere: al centrodestra e a quant'altri piacerebbe, probabilmente, disporre di forza lavoro senza pagare alcun prezzo da un punto di vista sociale, avere in sostanza a disposizione una casta di invisibili. Ma, rispetto alle trasformazioni ormai macroscopiche della società italiana ed europea, la politica rischia di rimanere un passo indietro: è necessario un progetto di ampio respiro, che guardi sì alla sicurezza, ma anche ai possibili modelli di integrazione che ormai investono aspetti economici, culturali e religiosi. Da qui non si esce. Essere padroni in casa propria non ha alcun senso, se quella casa e la nostra libertà di espressione sono minacciate. Più volte abbiamo auspicato che il primo articolo della nostra Costituzione possa essere riformulato in un'Italia fondata non tanto e non solo sul lavoro, ma sulla dignità della persona. È evidente che ogni cittadino deve poter agire liberamente, senza per questo sentirsi minacciato nella sua libertà d'espressione. Voglio ribadire che compito dello Stato è predisporre una serie di misure efficaci affinché il cittadino possa essere tutelato: in sintesi, non solo sia sicuro, ma soprattutto senta di esserlo, nell'adempimento dei doveri e nel rispetto delle regole. Ciò che evidentemente sfugge a queste «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» è che è la cultura della legalità a portare sicurezza, non viceversa.

Signor Presidente, osservo che nella politica italiana e nei percorsi parlamentari siamo diventati così raffinati e sofistici che siamo ormai oltre il dibattito sull'abuso e l'eccesso del ricorso al voto di fiducia, se è giustificato o no. Ormai siamo in grado di discutere e discettare di quale ricorso al voto di fiducia sia strumentale e inopportuno e di quale sia invece accettabile o rientri nella normalità dell'economia procedurale del percorso politico e parlamentare. Ebbene, a voler non adeguarsi, ma tuttavia prendere atto di questa estrema sofisticatezza nella quale ormai ci siamo avventurati, mi permetterei di dire che questo è un esempio di fiducia non abusata.

che è stato largamente dibattuto in tutti i circoli politici, perfino in una campagna elettorale e in molte sedi parlamentari, con particolare riferimento naturalmente all'altra Camera, quale, quindi, si è detto tutto e il contrario di tutto sul piano ideologico, sviscerandolo in tutte le sue articolazioni normative e tecniche. Detto questo, voglio anche aggiungere che devo constatare che la nostra opposizione dimostra veramente la sua incultura di governo. Mi dispiace usare questa espressione severa, ma è così. Di fronte ad un'opinione pubblica che spinge su tutti, su noi della maggioranza, del Popolo della libertà, così come sulle opposizioni di centrosinistra, perché qualche cosa di concreto, di incisivo, di percepibile, di efficace si faccia

colleghi senatori dell'Italia dei Valori usare un frasario e una cifra logica che francamente non avevo mai sentito usare nella sua assurdità e nel suo integralismo ideologico nemmeno dalla sinistra più estrema, in entrambe le Camere che ho avuto l'onore di frequentare. Quindi, vorrei dire che è tutta l'opposizione ad essere accecata in qualche modo dalla sua volontà di dire «no, no, no» a raffica, a tutti i provvedimenti che dalla maggioranza governativa vengono finisce per dimostrare palesemente all'opinione pubblica, che eventualmente ci stia ascoltando, la sua incultura di governo. Non fa dunque meraviglia se sempre più questa sinistra si distacca dall'opinione pubblica dai cittadini. E non varranno le diatribe congressuali, questo o quel personaggio, lenzuolate o non lenzuolate, i giri in treno di questo o quel presunto *leader* del Partito Democratico, quando si è in rotta frontale con le richieste fondamentali che il cittadino, l'uomo e la donna comune, anziani e giovani, fanno salire, molto spesso con un grido di dolore. Abbiamo sentito prima un collega della sinistra - seppure di una frazione del Gruppo del Partito Democratico, ma comunque facente parte di quel Gruppo - mettere addirittura in dubbio che vi sia un'emergenza e affermare che l'Italia, tutto sommato, è forse il Paese più sicuro dell'Occidente e dell'Europa. Ma come si possono dire queste cose, che suonano come una provocazione ad un'opinione pubblica e a dei cittadini che esigono da noi interventi concreti e reali?

ma non c'è un solo passaggio, un solo articolo sul quale, colleghi dell'opposizione, non abbiate detto un no, in profonda contraddizione anche con le vostre stesse premesse. Se è per voi, la conclusione ve la dico io qual è: non si deve far nulla. Le carceri sono affollate? Allora non bisogna adottare sanzioni penali, altrimenti si fa scoppiare una situazione. Non si riesce a disciplinare un certo flusso immigratorio sregolato che dà luogo a tanti problemi? Allora Allora apriamo semplicemente le frontiere e organizziamoci per l'accoglienza migliore. Si fanno provvedimenti che impongono misure d'integrazione reale da parte di colui che vuole immigrare regolarmente? No, sono prevaricazioni rispetto ai diritti civili e ai diritti umani. Non si può far niente; qualunque cosa si faccia siete contrari. Si coinvolgono i cittadini in forme pur lecite e controllate per collaborare con le forze dell'ordine alla sicurezza? No, si sta facendo squadrismo e si stanno facendo le ronde. Si vogliono mettere i militari, i nostri ragazzi e ragazze delle Forze armate, a coadiuvare nelle zone più calde e critiche perché si controlli e si prevenga? No, si sta militarizzando il Paese e si sta violando ogni sorta di regole sulla ripartizione delle competenze.

i regimi comunisti, ancora ce n'è qualche residuo ma comunque ce li ricordiamo nelle loro epoche d'oro: lì in merito al problema della sicurezza, statene pur certi, non si andava né per buonismi, né per garantismi, né per norme costituzionali; non ci si andava e non ci si va.

distanziandosi sempre di più da quel buonsenso assolutamente medio che ormai i cittadini, quand'anche in passato avessero votato per i vostri partiti, li richiama a dire: ma che ho fatto? *(Il microfono si

rappresentanti del Governo, il provvedimento di cui stiamo discutendo oggi, recante «Disposizioni in materia di sicurezza

come ricordato in una serie di documenti in materia di sicurezza stradale adottati dalla Commissione europea. Così pure si sa che tutti gli interventi intesi a prevenire o a sanzionare tali comportamenti di guida pericolosa sono considerati prioritari dalle istituzioni comunitarie anche al fine di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di dimezzare, entro il 2010, il numero delle vittime di incidenti stradali. Tuttavia, i problemi legati alla piena attuazione nel nostro Paese di una vera cultura della sicurezza, e segnatamente della sicurezza stradale, avvertita sempre più come un'emergenza sociale, richiedono, a nostro avviso, un intervento molto più deciso e articolato di quello contenuto in questo provvedimento. Attualmente la Commissione trasporti della Camera dei deputati sta esaminando, in sede legislativa, un corposo provvedimento che contiene numerosi interventi di modifica del codice della strada; provvedimento che mi auguro riesca ad analizzare quanto prima anche il Senato della Repubblica, perché quello della incidentalità stradale è un tema talmente serio che merita di essere esaminato in modo sicuramente urgente, ma anche in modo approfondito e appropriato. In ogni caso, il senso del messaggio che vorrei trasmettere al Governo, in questo momento è esattamente questo: non possiamo non possiamo continuare a trattare il problema della sicurezza stradale nel nostro Paese in maniera disorganica e frammentaria senza intervenire in modo strutturale e fortemente responsabile. Il forte impatto sull'opinione pubblica e sul mondo dell'informazione di incidenti che hanno destato grande clamore, unitamente agli interventi di medio periodo della Commissione europea, che ha avviato un programma d'azione sulla sicurezza stradale agli inizi del 2000, hanno determinato negli ultimi anni una serie di iniziative che tuttavia non hanno avuto la conseguenza di introdurre un sistema virtuoso nel quale le *performance* di sicurezza del Paese possano essere considerate acquisite, stabili ed autoalimentate. Inoltre, si sta diffondendo, in particolare tra i cittadini, l'esigenza di interventi efficaci e severi finalizzati a reprimere comportamenti rischiosi. Con riferimento al 2007 - secondo gli ultimi dati ufficiali ISTAT- il nostro Paese, infatti, pur avendo registrato un significativo decremento nel numero dei decessi, per cento, è stato purtroppo segnato da un decremento decisamente meno lieve in termini di riduzione del numero di feriti e incidenti, rispettivamente pari al 2,1 per Peraltro, sebbene l'obiettivo fissato dall'Unione europea sia quello di ridurre, entro il 2010, il numero delle vittime e dei feriti del 50 sappiamo già che il nostro Paese non riuscirà a raggiungerlo e questo non deve far dimenticare al Governo che l'Italia ha bisogno di nuovi interventi strutturali che siano in grado di migliorare ulteriormente la situazione, nonché la spesa sociale, tuttora elevata, che il fenomeno determina. Tra l'altro, l'Italia è in controtendenza rispetto ad altri Paesi, dove si assiste ad una certa stabilità nel numero di incidenti, anche in Stati nei quali negli anni scorsi si erano raggiunti decrementi significativi. Questo a dimostrazione che se l'attenzione rispetto alle politiche per la sicurezza si allenta, i miglioramenti raggiunti non possono essere considerati acquisiti una volta per tutte. I Paesi che sono più vicini all'obiettivo del 50 per cento in meno e che con ogni probabilità lo centreranno sono la Francia e il Portogallo; i più lontani sono i Paesi dell'Est. sono i Paesi dell'Est. L'Italia, con 87 morti per milione di abitanti, pur collocandosi in linea con la media europea, che è di 86 resta comunque ben al di sopra dei livelli delle Nazioni che vantano le migliori *performance*, quali Olanda, Regno Unito e Svezia, con 45-50 decessi per milione di abitanti, e della Francia, che ne conta 73. Inoltre, è utile segnalare che esiste, nel nostro Paese, una forte esposizione del mondo giovanile al rischio legato all'incidentalità stradale, sia in termini di incidenti (circa il 30 pei cento avviene nei primi 3 anni dopo il conseguimento della patente)

necessari a livello istituzionale che sia capace di coinvolgere organicamente tutti i Ministeri interessati e gli enti territoriali, ma soprattutto credo che permanga una cronica carenza di risorse, mentre si continua ad insistere con la logica dell'intervento *spot*, non coordinato, non sinergico e spesso attuato sulla scia emotiva di incidenti particolarmente eclatanti. Il Piano nazionale per la sicurezza stradale, principale strumento di programmazione, non è stato mai finanziato nel periodo 2004-2006. E non sono ancora disponibili le risorse stanziate nella legge finanziaria per il 2007 per il triennio 2007-2010. Con una simile carenza di risorse, nessun intervento strutturale potrà evidentemente essere intrapreso. Con la legge finanziaria per il 2008, il Governo Prodi aveva ritenuto necessario, oltre che opportuno, investire un congruo ammontare di risorse finanziarie al fine di implementare le azioni tese ad accrescere la sicurezza stradale e dare attuazione al piano nazionale, mediante interventi mirati e sinergici, volti a rafforzare i controlli, anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature tecniche; intensificare l'attività ispettiva e le verifiche previste dal codice della strada; dotare gli uffici ed il personale preposto ad attività di sicurezza stradale degli opportuni strumenti per l'esercizio delle attività istituzionali, ivi compresa la formazione. Purtroppo, con il decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008 il Governo Berlusconi ha operato un drastico ridimensionamento dì dette risorse finanziarie, dimezzando lo stanziamento per l'anno in corso e annullando quelli relativi agli anni 2009-2013, pari ad un taglio complessivo di 181,5 milioni di euro. di tali considerazioni, a nome del Gruppo dell'Italia dei Valori intendo chiedere al Governo in primo luogo di restituire le somme che, in modo responsabile, il centrosinistra guidato da Prodi aveva destinato alla sicurezza stradale, in secondo luogo di smetterla di intervenire su questo tema in modo perennemente disorganico e insufficiente, anche al fine di non vanificare la possibilità che nel nostro Paese vengano create le condizioni materiali ed organizzative per contribuire alla riduzione del tragico bilancio della sinistrosità stradale, in coerenza - come già sottolineato - con gli obiettivi dettati dall'Unione europea. infine, che il costo dell'incidentalità stradale è di oltre 30 miliardi di euro ogni anno, pari a due punti percentuali del PIL. Questo significa che un miglioramento dell'incidentalità del 10 per cento permetterebbe di risparmiare 3 miliardi di euro ogni anno. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi senatori, c'è chi tenta di utilizzare l'assistenza ai minori (doverosa) come cavallo di Troia per scardinare il sistema delle regole sull'immigrazione. Non posso allora non ricordare che i dati ufficiali dicono che ci si integra con minori difficoltà dove si ha invece il coraggio di abbandonare il buonismo e si impongono regole precise. Tanto che ai primi posti per qualità dell'integrazione troviamo località come Treviso e Verona, amministrate dalla Lega Nord. Lo stesso cardinale Bagnasco, arcivescovo di Genova (città che ha i suoi problemi per la forte presenza di immigrati), riconosce che bisogna coniugare all'accoglienza «un altro principio, non meno necessario, quello della legalità, di cui tutti» - afferma - «si avverte la necessità per la convivenza sociale». Oggi la crisi economica ha ridotto i posti di lavoro, mentre la pressione migratoria verso i nostri confini non è mai stata così forte e organizzata. La percentuale di stranieri fra i denunciati e condannati per reati come borseggio, furto in appartamento, scippo, rapina, traffico di droga, stupro, omicidio è in costante crescita.

dati impongono un controllo capillare del territorio (se serve anche con le ronde, spinte dal senso civico, un tempo patrimonio di tutta la comunità), certezza delle pene e di rendere rapido ed efficace il sistema delle espulsioni. Gli altri Paesi offrono un ventaglio di soluzioni. La Spagna, ad esempio, dal 2000 ha stabilito una rigida programmazione dei flussi, prevedendo sanzioni per chi favorisce l'immigrazione clandestina (compresi i datori di lavoro che assumono in nero), oltre all'immediata espulsione degli stranieri residenti illegalmente. Per entrare nel territorio spagnolo servono tre requisiti: il possesso di documenti validi di identità, la prova di avere sufficienti mezzi di sostentamento per la durata del soggiorno e la prova dello scopo e delle condizioni del soggiorno. La cittadinanza può essere richiesta solo dopo dieci anni di residenza e non prima del diciottesimo anno di età. In Francia, una legge del 2003, che porta la firma dell'attuale presidente Nicolas Sarkozy, ha introdotto un'attenta regolamentazione degli ingressi. La lotta all'immigrazione clandestina è stata rafforzata attraverso molteplici misure: dalla schedatura di coloro che fanno richiesta di visti o permessi di soggiorno attraverso impronte digitali e dati biometrici, all'inasprimento delle pene per i trafficanti di esseri umani. La carta di residenza viene accordata dopo cinque anni: requisito fondamentale per ottenerla è la conoscenza della lingua transalpina e dei princìpi della Repubblica francese. Il Regno Unito ha introdotto una politica migratoria indirizzata ai lavoratori qualificati. Gli altri vengono invece scoraggiati. Esiste infatti un sistema a punti: secondo l'età, la situazione finanziaria, il livello di istruzione, le eventuali qualifiche e la conoscenza della lingua inglese. C'è poi l'obbligo - che decade solo per gli iperqualificati - di presentare un certificato di sponsorizzazione da parte di un datore di lavoro o di un istituto scolastico. Sulla stessa linea è la Germania che, con quasi sette milioni di immigrati, è il più grande Paese d'immigrazione in Europa. Dal 2005 ha avviato una politica d'incoraggiamento dell'immigrazione qualificata, che consente di ottenere la residenza e il permesso di lavoro fin dall'inizio. Requisito essenziale è avere una concreta offerta di lavoro e il permesso dall'Agenzia tedesca per l'impiego. I clandestini possono essere detenuti per garantire la loro effettiva espulsioneper sei mesi prorogabili C'è poi il codice americano, che prevede il reato di «entrata impropria di straniero», violazione della «legge civile e penale», punibile con multe o con il carcere fino a sei mesi, e fino a due anni in caso di comportamento reiterato. A parte, abbiamo un reato di reingresso illegale, nel quale incorre chi è sorpreso a tentare di entrare negli USA dopo avervi commesso reati. Ma meno del 4 per cento del milione di arrestati finisce sotto processo.

Con la Lega Nord al Governo, l'Italia prova ad affrontare in modo innovativo la questione dei rimpatri di clandestini, diventati complicati e costosi. Inizia l'era dei respingimenti. D'ora in poi, una volta intercettati, i migranti delle carrette del mare dirette verso le nostre coste saranno respinti prima di entrare in acque nazionali e riportati nel luogo di partenza. La nuova strategia è stata inaugurata con lo stop a tre barconi, restituiti subito ai porti della Libia. Risultato: il flusso si è fermato; i migranti non rischiano più la vita in mare. Per quanto riguarda il trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione, nei palazzi romani si è discusso a lungo sull'opportunità di trattenere i clandestini nei CIE oltre i sessanta giorni previsti dalla nostra normativa, quando necessario per completare l'*iter*, come chiesto dal ministro Maroni. Ma è la stessa Unione europea a dire che «si può trattenere lo straniero» sottoposto a procedura di rimpatrio se lo stesso ostacola il procedimento di identificazione e che «ogni Stato stabilisce il suo periodo di trattenimento, che in ogni caso non può superare i sei mesi». È possibile raggiungere i dodici mesi «nei casi in cui, nonostante siano stati compiuti tutti gli sforzi che è lecito aspettarsi, l'operazione dell'allontanamento rischia di prolungarsi più a lungo a causa della mancata collaborazione da parte del clandestino o dei ritardi nell'ottenimento dei necessari documenti da parte del Paese terzo». In casi particolari, senza collaborazione dello straniero si può arrivare addirittura a diciotto mesi di trattenimento. È meno chiara l'Unione europea sui rimpatri. È infatti prevista l'emissione del cosiddetto foglio di via, con un termine per la «partenza volontaria» dell'irregolare fra i sette e i trenta giorni, sistematicamente ignorato. Da qui la nostra richiesta d'introdurre il reato di «ingresso e permanenza illegale nel territorio dello Stato» - già presente in molti Paesi - sanzionabile con un'ammenda (per non sovraffollare le carceri) e l'espulsione effettiva come pena accessoria. *(Applausi

al 27 per cento. Desidero al riguardo rassicurare l'Assemblea che la Presidenza ha già richiamato su tale questione l'attenzione del Governo, al quale ha rivolto un invito a corrispondere in tempi brevi ai documenti di sindacato ispettivo in attesa di risposta. Per offrire un elemento di raffronto, si segnala che anche nella precedente legislatura si è registrata una tendenza analoga. Infatti, a distanza di un anno dall'avvio della XV legislatura,